la ricerca*. In merito al caso dell'alunna cui si fa riferimento nell'atto in discussione, è stata interessata la competente direzione scolastica regionale per la Toscana che, al riguardo, ha riferito quanto segue. Lo scorso 9 dicembre su alcuni quotidiani («Il Giornale della Toscana», «la Repubblica», «La Nazione») sono apparsi articoli che evidenziavano il caso di una quindicenne musulmana frequentante la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo statale di Reggello, in provincia di Firenze, Firenze, costretta a tapparsi le orecchie con delle cuffie durante la lezione di musica, a quanto si apprendeva, per volontà del padre, per il quale l'ortodossia religiosa musulmana vieterebbe l'ascolto della musica. Appresa la notizia, l'ufficio scolastico regionale ha immediatamente disposto, il 10 dicembre, visita ispettiva *in loco* da parte di un dirigente tecnico. Gli accertamenti ispettivi hanno confermato le notizie apparse sulla stampa. Sul piano strettamente didattico, è stato evidenziato che il percorso personalizzato di educazione musicale predisposto per l'alunna in parola confliggeva con quanto previsto dall'ordinamento scolastico, perché andava a ridurre una parte degli obiettivi di apprendimento previsti dalle indicazioni della scuola secondaria di primo grado per questa disciplina. Il giorno successivo, 11 dicembre, è stato convocato a scuola il padre dell'alunna per metterlo a conoscenza del fatto che la situazione scolastica della figlia andava riesaminata perché incompatibile con l'ordinamento scolastico vigente. Dopo il colloquio con il competente dirigente scolastico, il padre dell'alunna è apparso più conciliante e disposto a rivedere la propria posizione. Si è avuto, altresì, un colloquio anche con l'alunna per convincerla a rinunciare alle cuffie e ad entrare nell'aula di musica mentre i compagni suonavano, cosa che è avvenuta il 13 dicembre, data dalla quale l'alunna è in classe senza l'utilizzo delle cuffie. Da tale data, quindi, l'alunna segue regolarmente le lezioni pratiche di educazione musicale senza il ricorso al detto mezzo di isolamento. La positiva e rapida conclusione della vicenda si è resa possibile, da un lato, grazie all'immediato intervento ispettivo dell'ufficio scolastico regionale e, dall'altro, grazie al forte e deciso coinvolgimento della famiglia dell'alunna da parte delle componenti scolastiche interessate.

nell'interrogazione che noi abbiamo presentato immediatamente dopo la notizia, sollevando il caso, oltre al tema specifico, volevamo riportare l'attenzione del Governo e degli organi che vigilano sulla scuola

la questione principale sollevata nell'atto in discussione concerne il riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio di insegnamento non di ruolo prestato nelle scuole paritarie private. A tale proposito, nell'interrogazione viene rilevato che la mancata valutazione del servizio in esame, in relazione al diverso trattamento dei servizi prestati nelle istituzioni scolastiche statali, non sarebbe giustificata in quanto anche le scuole paritarie fanno parte del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge n. 62 del 10 marzo 2000 sulla parità scolastica. Va premesso che le fattispecie dei servizi riconoscibili ai fini della carriera sono tassativamente individuate per legge e non sono quindi possibili interpretazioni estensive della norma che, come nel caso prospettato, comporterebbero riflessi finanziari. Considerato che la legge n. 62 del 2000 non contiene alcuna espressa previsione al riguardo, la materia è tuttora disciplinata dal decreto legislativo n. 297 del 1994 - articolo 485, commi 1 e 3 - in base al quale, come è noto, il servizio prestato presso le scuole statali, pareggiate e parificate è riconosciuto come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici per intero per i primi quattro anni e per i due terzi per il periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. Il problema sollevato non può pertanto trovare soluzione in via amministrativa. Quanto, poi, all'ulteriore questione segnalata, concernente il trattamento economico del personale docente assunto nelle scuole paritarie private, esula dalla competenza di questa amministrazione ogni valutazione sui contenuti dei contratti collettivi di lavoro che le associazioni di gestori privati sottoscrivono con le organizzazioni sindacali.

e cioè che il servizio prestato presso queste scuole è riconosciuto come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici per intero per i primi quattro anni e per i due terzi per il periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il restante terzo. Ciò non avviene, signor Sottosegretario, e non per colpa della contrattazione nazionale, ma dell'amministrazione, perché c'è una legge dello Stato che sancisce come deve essere regolata la materia,

Signora Presidente, l'istituto del riscatto dei corsi universitari di studio, previsto dalla legge n. 114 del 1974 ed esteso agli iscritti alla gestione separata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. del 1997, si applica ai corsi al termine dei quali siano stati ottenuti i diplomi previsti dalla legge n. 341 del 1990, ossia il diploma universitario, il diploma di laurea, il diploma di specializzazione ed il dottorato di ricerca. Le leggi nn. 508 del 1999 e 268 del 2002 hanno introdotto una riforma degli istituti artistici e hanno dettato misure urgenti per l'impiego dei relativi titoli stabilendone l'equipollenza alle lauree di cui al decreto ministeriale 509 del 1999 con lo specifico fine dell'accesso ai pubblici concorsi e sempre che i titoli siano stati conseguiti da soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di formazione artistica e musicale, sono stati attivati presso gli istituti AFAM nuovi percorsi didattici a decorrere dall'anno accademico 2005-2006, che danno luogo al conseguimento di appositi titoli di studio. In relazione a tale regolamento, il Ministero, con nota protocollo n. 4172 del 4 giugno 2008 ha chiarito che «gli studenti del Presidente della Repubblica n. 212/2005 hanno diritto alle stesse provvidenze destinate agli studenti universitari», sostenendo così la necessità di ammettere a riscatto i titoli in parola sulla base delle argomentazioni giuridiche riportate dall'interrogante. Il problema del riscatto dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni del sistema AFAM è stato oggetto di una fitta corrispondenza tra la direzione generale AFAM, gli enti previdenziali interessati (INPS ed INPDAP) e il Ministero del lavoro ed altresì di appositi tavoli tecnici sviluppatisi fino al mese di aprile dello scorso anno. Dalla citata corrispondenza, nei vari anni è emersa una posizione netta dell'INPDAP, da ultimo espressa in via generale con nota operativa 25 del 14 maggio 2009, per cui l'ente ammette a riscatto esclusivamente gli anni a decorrere dall'anno accademico 2005-2006, in ottemperanza all'entrata in vigore del regolamento didattico ed in particolare dell'articolo 3 del decreto del L'INPS, che in un primo approccio sembrava essere più possibilista, non ha ritenuto opportuno, allo stato dei fatti, discostarsi dalle determinazioni assunte dall'INPDAP e si è espressa sulla questione con il messaggio n. 015662 del 2010, ammettendo a riscatto i nuovi corsi attivati a decorrere dall'anno accademico 2005-2006 che diano luogo ai titoli previsti dal citato regolamento tuttavia, assumendo che i diplomi accademici conseguiti in base all'ordinamento previgente continuano ad essere equiparati ai diplomi di laurea (unitamente al possesso di un titolo di scuola superiore) solo ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, con ciò escludendone una equiparazione in termini assoluti ed in particolare ai fini del riscatto contributivo. Nello specifico caso prospettato dall'interrogante, alla luce delle considerazioni svolte, l'INPS ritiene che la competente direzione provinciale, nel respingere la domanda di riscatto, abbia correttamente applicato le disposizioni impartite con il suddetto messaggio, trattandosi di un titolo conseguito al termine di un corso di studi iniziato prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, privo quindi della menzionata equiparazione. Sul fronte giurisprudenziale è, comunque, opportuno rilevare che, in relazione alla questione in esame, l'INPS è già risultata soccombente, sia in primo grado che in appello, ed è stata altresì condannata alla liquidazione delle spese (sentenza della corte di appello di Torino - sezione lavoro 1429 del 2007). In base alle argomentazioni a sostegno della sentenza è plausibile sostenere che ogni altra azione giudiziale venisse in tal senso intrapresa avrebbe uguale risultato. Si deve, inoltre, rilevare che, per quanto riguarda i diplomi delle Accademie di belle arti, la Corte costituzionale, già con le sentenze n. 535 del 1990 e n. 52 del 2000, aveva riconosciuto riscattabile il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l'Accademia di belle arti, ciò quando il relativo diploma o titolo di studio fosse richiesto come *condicio sine qua non* per l'accesso ad un pubblico impiego.

Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, e ciò nella prevalente considerazione dell'avvenuta equiparazione, a decorrere dall'anno accademico 2005-2006, fra l'iscrizione agli istituti di alta formazione artistica e musicale e l'iscrizione ai corsi universitari».

possano pesare dal punto di vista dell'interpretazione giuridica, mi permetto di definirmi abbastanza soddisfatta. Come minimo, da parte sua e del Governo vi è stata la ricognizione di un *excursus* piuttosto complicato e articolato, che in questi anni ha visto le istituzioni che riguardano l'alta formazione artistica e musicale, vale a dire accademie, conservatori

questa equiparazione, così sofferta (portai avanti personalmente questa battaglia), era un atto dovuto, perché in ogni Paese europeo e del mondo coloro che frequentano accademie e conservatori hanno un titolo di studi che corrisponde alla laurea; nei concorsi internazionali per le grandi orchestre, per le grandi mostre artistiche, i nostri studenti non venivano ammessi perché il titolo, benché avessero il diploma di istruzione secondaria superiore, non era equiparato ad una laurea, laurea, era considerato un diploma. Quindi, nonostante gli stranieri vengano a studiare da noi, si formino ai nostri conservatori, alle nostre accademie, che hanno un profilo altissimo, di eccellenza, per quanto riguarda la didattica e la capacità operativa a livello artistico, noi noi avevamo i nostri studenti impossibilitati a partecipare ai concorsi internazionali. Fu una grandissima battaglia: una battaglia di civiltà, una battaglia di giustizia, vinta e poi naturalmente caduta nel dimenticatoio per responsabilità politica fortissima dei Governi che si sono succeduti che non hanno dato attuazione concreta a quella legge. Ad oggi qui, in Senato, abbiamo delle proposte proposte di riforma per mettere fine al contenzioso, ma si cincischia continuamente, avvitando le procedura, le note legislative, i messaggi - come lei ha detto - anche da parte di istituzioni esterne allo Stato, che

sul come stanno morendo l'arte e la cultura italiana nell'alta formazione artistica, prive di quattrini, messe in una sorta di limbo dove non si sa che fine faranno, a cui bisogna dare una risposta. Questo Governo si fa vanto della capacità di valutare e valorizzare il merito e l'eccellenza. Quale migliore eccellenza oggi nel mondo possiamo presentare se non quella, ancora, dei nostri beni culturali, del settore artistico e dell'alta formazione, dove ancora siamo capaci di competere grazie all'intelligenza, alla forza creativa dell'intelligenza e della sensibilità dei nostri giovani studenti? Per quale motivo non si mette mano a

perché questo settore sta morendo. Facciamoci carico di tale operazione, altrimenti poi non piangiamo se cadono le rovine storiche di Pompei o i monumenti. Qui cadono anche gli animi, le intelligenze, le sensibilità, frustrate da un sistema che non le comprende, non le sostiene e soprattutto non incentiva assolutamente un percorso di approfondimento e di creatività di cui abbiamo assolutamente bisogno, perché è la nostra vera, unica materia prima.

e alla scuola paritaria. Il principio costituzionale della libertà di educazione trova realizzazione, oltre che attraverso le scuole statali, anche tramite le scuole non statali riconosciute paritarie ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62. È necessario quindi dare risposte adeguate alle esigenze di istruzione e formazione del cittadino, mediante la realizzazione di un sistema pubblico che fondi sul principio di sussidiarietà forme di pluralismo educativo, per garantire agli studenti una scuola di qualità, in linea con gli standard europei ed internazionali, indipendentemente dal fatto che sia statale o privata paritaria. Le scuole paritarie, pertanto, siano esse confessionali, laiche o espressione degli enti locali, fanno parte integrante del sistema nazionale di istruzione e i fondi statali, previsti con la legge di stabilità, tra l'altro ampiamente condivisi in seno parlamentare, sono erogati al fine di sostenerne la funzione pubblica. Il riconoscimento della parità scolastica impegna, peraltro, le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola. L'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, istitutiva della scuola paritaria, al proposito, specifica al comma 1: «Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita». Per quanto riguarda i finanziamenti scolastici c'è da osservare che la legge n. 244 del 2007 prevedeva economie di spesa pari ad euro 535 milioni per il 2008; 897 milioni per il 2009; 1.218 milioni 1.218 milioni per il 2010 ed euro 1.432 milioni per il 2011, senza che vi fossero interventi ordinamentali di riforma del sistema scolastico. Successivamente, la legge n. 133 del 2008 ha delegato il Governo a riformare il sistema scolastico, al fine di allinearne i parametri al sistema europeo, sia in termini di offerta formativa che di rapporto nel numero docenti-studenti. A tal fine, l'articolo 64, comma 6, della legge n. 133, prevede economie di spesa pari a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 3.188 milioni per l'anno 2012. Complessivamente, a regime, dal 2012, le economie di spesa risulteranno quindi pari a 4.620 milioni di euro all'anno, cifra che non corrisponde ad 8 miliardi di euro come sostenuto nell'interrogazione. In un momento delicato, come opportunamente si sottolinea anche in questa interrogazione parlamentare, il Governo ha dimostrato la dovuta attenzione al grave problema della retrocessione della qualità del nostro sistema formativo scolastico e universitario, che ha radici chiaramente antiche, rispetto agli altri Paesi dell'Unione Europea. Si sta perciò facendo ogni necessario sforzo, dimostrando nei fatti concreti di voler tenere conto, nonostante i problemi che interessano il pianeta scuola, degli impegni assunti nel Vertice di Lisbona e per dare, come opportunamente richiamato nell'atto in questione dalla senatrice, nuovo impulso alla qualità didattica e all'organizzazione gestionale della scuola pubblica statale. Per la prima volta dal 1923, l'anno scolastico è iniziato appunto con una riforma ordinamentale compiuta e completata in tutti i cicli scolastici e con l'avvio della messa a regime del sistema di istruzione, nonché del sistema di istruzione e formazione professionale, affidato alle Regioni. È attiva infatti, a partire dalle prime classi del nuovo anno scolastico 2010-2011, la riforma della scuola secondaria superiore. Con il 1° settembre sono stati avviati i nuovi licei, i nuovi istituti tecnici e i nuovi istituti professionali. Un provvedimento innovativo che riduce infatti la frammentazione degli indirizzi nei licei e rilancia l'istruzione tecnica e professionale. Il settore tecnico-scientifico è stato al centro dei principali cambiamenti introdotti con la riforma che, come dimostrano i dati sulle iscrizioni, hanno riscontrato il favore degli studenti e delle famiglie. Rispetto all'anno precedente l'aumento delle iscrizioni in questo settore è dell' 1,7 Per quanto riguarda la scuola primaria, aumentano le classi a tempo pieno. In questo nuovo anno scolastico sono passate da 36.493 a 37.275. Qualità e modernizzazione sono le parole chiave che caratterizzano lo spirito di questa riforma. Una scuola nuova al passo con i tempi, in cui si privilegia la qualità dell'insegnamento rispetto alla quantità del carico orario e all'eccessivo numero di materie, come raccomandato dall'OCSE. La stessa organizzazione internazionale, proprio nell'ultima parte del 2010, ha reso noti i risultati dell'indagine PISA (*Programme for international student assessment*) svolta nell'aprile 2009. Il rapporto segnala un grande successo dell'Italia che risale nelle classifiche europee di sei posizioni nella comprensione dell'italiano rispetto al 2006, di tre nella matematica e di una nelle scienze. L'Italia è dunque tra i Paesi che migliora maggiormente nella qualità scolastica a livello mondiale, come riconosciuto recentemente dall'OCSE. È un risultato questo apprezzato da tutti, al di là delle collocazioni politiche, perché permette all'Italia di invertire finalmente il *trend* negativo che durava da molti anni. Le classifiche internazionali mettono infatti il nostro Paese tra quelli che hanno avuto i più significativi miglioramenti. Per quanto riguarda la riforma universitaria, nonostante la crisi finanziaria, la stessa ha tracciato linee innovative, recuperato risorse significative, anche se non esaustive, e soddisfatto gran parte delle legittime richieste in campo. Per la prima volta, dopo anni di dibattiti, si è passati dai proclami, che spesso lasciano tutto fermo e statico, alla reale volontà di avviare un processo che ci consentirà di entrare da protagonisti nei grandi cambiamenti, che sono alla base del futuro economico-sociale e culturale del nostro Paese e della stessa Europa.

destabilizzante nei confronti del sistema dell'istruzione pubblica a livello primario, secondario ed universitario per favorire un sistema di tipo privatistico, come accade in altri Paesi. Noi non abbiamo la cultura, né la struttura sociale e politica per reggere a questo tipo di impatto. Se vogliamo che la massa di persone non acculturate sia sempre più ampia affinché in maniera più efficace si possa governare a proprio piacere e a proprio comodo, modo migliore è quello di destrutturare la scuola pubblica facendole mancare l'ossigeno e quindi i dovuti finanziamenti; nel contempo, si favoriscono le scuole private, là dove le regole valgono fino ad un certo punto, c'è una manica più larga, vi sono maggiori possibilità opzionali rispetto all'organizzazione e al funzionamento e, quindi, vi sono determinate garanzie (penso, ad

sistemi ed i metodi, però, sono tanti, dalla formazione continua dei docenti ad un impegno diverso, da una modernizzazione ad una ristrutturazione ordinamentale. Il problema è che manca l'ossigeno, vale a dire l'adeguato finanziamento, tanto che i nostri studenti, giovani e meno giovani,

determinato livello di istruzione e di formazione. Credo che effettivamente si debba ribilanciare e tarare la bilancia sulla Costituzione italiana, la quale non vale solo quando ci piace e ci pare, ma vale soprattutto per quello che vi è scritto, fintantoché vi sarà scritto. che le istituzioni private possono vivere e sopravvivere, essere competitive, purché non comportino oneri per lo Stato. Il ministro Tremonti ha prima tolto e poi ha

un certo settore per far dimenticare alcune manchevolezze del nostro *Premier*. Non è bello e non è giusto che i nostri studenti delle scuole pubbliche si vedano detratti i finanziamenti loro dovuti. I cittadini che pagano le tasse vogliono avere adeguati servizi e non con funzionamento ridotto. quindi avere gli stessi diritti che hanno tutti gli altri: prima la scuola pubblica, prima il servizio pubblico anche integrato, e poi le scuole private. Deve essere questo un motivo dominante nella cultura anche politica di un Governo che si dichiara liberale. Liberalità vuol dire vuol dire soprattutto pensare ad una istruzione di base alta per tutti, nella quale poi i migliori hanno la possibilità di accedere anche ai più alti livelli della formazione. Mi auguro che il Governo faccia una riflessione al riguardo e che simili comportamenti del Ministro dell'economia non vengano reiterati.

Mi riferisco all'interrogazione dei senatori Massidda e Sbarbati relativa al rinvenimento di alcuni reperti archeologici di estremo interesse scientifico, annunciato nel corso di una trasmissione televisiva dell'emittente sarda Videolina. Ritengo opportuno procedere iniziando dalla notizia relativa al vaso rinvenuto in località Arzachena, recante una "misteriosa scrittura", per sottolineare l'assoluta infondatezza del suo contenuto. Infatti il servizio, firmato dal giornalista Andrea Busia, faceva riferimento ad un vaso ritrovato durante una delle campagne di scavo dirette dalla dottoressa Angela Antona dal 2003 al 2008. In particolare, si tratta di un'olla con decorazioni plastiche fino ad allora inedite, rinvenuta in frammenti in un edificio (la "Capanna delle riunioni") del villaggio circostante il nuraghe La Prisgiona) in regione Capichera di Arzachena, e ricomposta durante le operazioni di restauro dei materiali. Del ritrovamento di tale reperto e dello studio del medesimo sono state date immediatamente e a più riprese notizie, corredate di foto e disegni, in contesti scientifici accreditati. La nutrita bibliografia che gli uffici mi hanno allegato dà chiaro riscontro dell'importanza attribuita al pezzo e della pronta risposta scientifica che ha suscitato negli uffici istituzionalmente deputati alla sua conservazione, tutela e valorizzazione. Non ci si è inoltre risparmiati sulla divulgazione, intervenendo in servizi televisivi nei quali sono state mandate in onda, insieme alle immagini del villaggio, quelle del vaso in questione (conferenza stampa organizzata sul sito nel maggio 2007 alla presenza di tutte le testate giornalistiche e televisive sarde), in conferenze organizzate in occasione delle Giornate europee

Università del tempo libero di Olbia), o con articoli in riviste di ampia diffusione. In relazione al frammento fittile da Pozzomaggiore Pozzomaggiore si precisa quanto segue. Il nuraghe Alvu di Pozzomaggiore è stato oggetto di un intervento di restauro e scavo archeologico nell'ambito del progetto «Il nuraghe Alvu tra fruizione e salvaguardia», con finanziamento della Regione Sardegna, dal novembre 2006 fino al dicembre 2007. I lavori, diretti dalla Soprintendenza per i beni archeologici per le Province di Sassari e Nuoro, hanno permesso di mettere in luce uno dei complessi monumentali nuragici più interessanti della Sardegna settentrionale e di evidenziare un'importante stratigrafia all'interno del complesso. Un ulteriore finanziamento da parte del Comune di Pozzomaggiore ha consentito di procedere con la documentazione grafica, ancora in corso, di tutti i reperti. Il frammento è attualmente conservato presso il centro di restauro della Soprintendenza archeologica delle Province di Sassari e Nuoro. Si procederà con la pubblicazione integrale dei risultati dello scavo dopo gli interventi di restauro. Una comunicazione sui risultati dell'indagine è stata presentata dagli archeologi Luisanna Usai e Franco Campus al convegno dell'Istituto italiano di preistoria e protostoria che si è tenuto a Cagliari nel novembre 2009. Gli stessi studiosi hanno presentato al comitato scientifico il testo per gli atti. Tutti gli ambienti scavati, ed in particolare il cortile, hanno permesso di evidenziare una sequenza stratigrafica che documenta, oltre alla fase nuragica, l'occupazione del nuraghe in età punica e romana, con sporadiche frequentazioni anche in età fenicia. Il reperto citato nell'interrogazione è chiaramente riferibile alle fasi di rioccupazione del nuraghe ed i caratteri della scrittura sono facilmente ascrivibili ad ambito fenicio-punico; ciò non contrasta neanche con la posizione stratigrafica del reperto. Per quanto riguarda la Navicella nuragica fìttile da Teti, devo riferire che l'immagine trasmessa dai promotori della petizione è risultata assolutamente incomprensibile agli archeologi delle nostre Soprintendenze che, d'altra parte,

come ben esplicitato in tutti i testi scientifici sulla civiltà nuragica, questa non ha mai conosciuto la scrittura. Del frammento proveniente da Villanovafranca o Senorbi gli uffici competenti dispongono della fotocopia di una fotografia. Sono in corso ricerche in proposito. Concludo sottolineando come il Ministero, nonostante i gravi tagli subiti, che incidono, soprattutto, sulla possibilità degli ispettori archeologi di presidiare il territorio, approntano sempre ed in tempi brevissimi sia il restauro che lo studio e la pubblicazione dei reperti ritrovati nel corso di scavi regolari.

veniva detto soprattutto in Sardegna su tali questioni. È bene essere precisi, anche culturalmente, rispetto a ciò che è stato ritrovato, al suo valore, ai tempi a cui può essere riferito e alla valenza che può avere anche come ricchezza di patrimonio da tutelare e conservare.

culturali*. Mi riferisco alle interrogazioni dei senatori Tomaselli, Della Seta e Ferrante, relative al giudizio favorevole espresso, per quanto di competenza, dal Ministero per i beni e le attività culturali, circa la compatibilità ambientale di un progetto presentato dalla società "Northern Petroleum" al fine di compiere indagini sismiche finalizzate alla ricerca di idrocarburi da realizzarsi al largo delle coste della Regione Puglia. Preciso, al riguardo, che la competente direzione generale, al fine di effettuare una compiuta valutazione dell'istanza, ha richiesto che la stessa società inviasse una copia cartacea e digitale del progetto a ciascuno dei propri uffici periferici. La Soprintendenza archeologica, nell'ambito della propria competenza e limitatamente alla prima fase del progetto, non ha ravvisato nel sistema di rilevamento geofisico prescelto alcun particolare pericolo di danneggiamento di eventuali relitti presenti sul fondo marino. Sottolineo «limitatamente alla prima fase del progetto», perché la stessa Soprintendenza ha evidenziato l'eventuale situazione di rischio nella seconda fase del progetto. Ad analoghe considerazioni sono addivenute la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto e la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Bari e Foggia, che hanno ritenuto i lavori previsti privi privi di effetti negativi nel contesto paesistico del sito, ma suscettibili di incidere su un tratto costiero di rilevante interesse paesaggistico qualora, in una seconda fase del programma di lavoro, si fosse programmata l'installazione di strutture metalliche fisse. La competenza del Ministero per i beni e le attività culturali si esaurisce, come noto, in questi adempimenti, preposti alla conservazione ed alla tutela paesaggistica ed archeologica dei siti oggetto dell'intervento, dal momento che, si rammenta, lo studio di impatto ambientale andava riferito alla prima fase del Programma L'amministrazione tuttavia, consapevole del delicato equilibrio ambientale della zona, ne ha rammentato, nel proprio provvedimento, il valore e l'esigenza di salvaguardia. Inoltre il direttore generale, nell'esprimere il suo parere, peraltro sottoposto alle condizioni che la Soprintendenza archeologica aveva inteso dettare, anticipava, nell'ipotesi dell'avvio di una seconda fase, la necessità che per essa si presentasse

deliberazioni delle vostre strutture periferiche, se così possiamo chiamare le Sovrintendenze, che agli interroganti erano note, e infatti erano oggetto della nostra preoccupazione nelle interrogazioni. Il punto per cui non possiamo

ambientale - mi limito a leggere testualmente l'ordinanza - «rilevato che il procedimento di compatibilità ambientale è culminato nella adozione di provvedimenti ministeriali che sembrano avere disatteso alcuni considerevoli profili di criticità qui di seguito riportati: omesso perfezionamento della procedura di composizione della commissione tecnica di verifica di impatto ambientale mercé convocazione del rappresentante designato dalla Regione Puglia, con conseguente mancata valutazione di interessi ascrivibili all'ente territoriale; omessa considerazione del carattere inquinante della tecnica di prospezione geofisica denominata "Air Gun", soprattutto in rapporto alla mancata considerazione di un'alternativa tecnicamente praticabile allo stato delle conoscenze di settore e delle caratteristiche di sensibilità dell'area non adeguata considerazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dall'utilizzo della suddetta metodica di prospezione geofisica per la salvaguardia di alcune specie marine

locali, l'aver dato, in assenza di queste specifiche, l'autorizzazione ad una società petrolifera per andare a cercare petrolio, che peraltro molte indagini ci dicono essere di bassa qualità. Quindi bisogna anche valutare per il sistema Paese se vale la pena correre questo rischio. Non voglio qui ricordare disastri ambientali avvenuti in questo ultimo periodo

facendo un regalo ad un'azienda petrolifera straniera che può utilizzare metodiche poco rispettose del territorio e dell'ambiente. conclusione, ci permetteremo di reiterare la nostra richiesta fin quando sarà il Ministero dell'ambiente a rispondere in maniera più completa di quanto lei oggi ha potuto fare alle nostre preoccupazioni.